questa mattina sulla tratta Corato-Andria delle Ferrovie del Nord Barese si è verificato un gravissimo incidente tra due convogli che viaggiavano in direzione opposta su un binario unico. Le prime notizie che giungono dal luogo del disastro danno il quadro di una tragedia di proporzioni terribili. Secondo un primo bilancio, ancora provvisorio, ci sarebbero almeno 20 morti e diverse decine di feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. Le immagini mostrano vagoni sbriciolati nell'impatto, pezzi di lamiere volati per decine di metri nella campagna ai lati dei binari su una linea ferroviaria utilizzata soprattutto da studenti e lavoratori pendolari. Una volta conclusa l'opera di soccorso sarà necessario fare chiarezza sulle dinamiche e le cause dell'incidente in modo da evitare che tragedie come questa possano ancora ripetersi. Alle vittime di questa sciagura va il pensiero commosso del Senato, unito al cordoglio per le famiglie, ai feriti l'augurio di un pronto ristabilimento, a tutti coloro che si stanno prodigando nell'opera di soccorso il nostro convinto ringraziamento. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.

i comunicati stampa si sono susseguiti con ritmo incessante, fino a diventare veri e propri bollettini di guerra, bollettini di guerra, che hanno trasformato il territorio della mia Regione compreso tra Andria e Corato

per commentare l'accaduto e riportare gli aspetti di una vera e propria tragedia, una tragedia di proporzioni incredibili che ci è stata consegnata con immagini di una vera e propria apocalisse: due treni che si sono scontrati percorrendo un unico binario ad una velocità elevata. non è questo il momento per allungare il dito indice accusando nessuno. Questo è il momento di esprimere la nostra profonda vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i propri congiunti, a tutte le famiglie che hanno, in queste ore, il cuore tribolante per le condizioni dei feriti feriti e credo che, accanto a questo pensiero, vada aggiunta anche una nota di apprezzamento per la mobilitazione generosa di tutte le forze di volontariato e per l'organizzazione puntuale e tempestiva dei servizi sanitari del territorio, che sono giunti sul luogo della tragedia per prestare i soccorsi con efficienza e tempestività. dobbiamo necessariamente rinviare a tempi brevissimi un approfondimento sulle motivazioni che hanno determinato questa tragedia, in una Regione che resta assolutamente marginalizzata a causa del *gap* infrastrutturale che la penalizza.

inconsapevoli di andare invece incontro alla morte. Signor Presidente, la ringrazio per aver dedicato un momento di attenzione a questa tragedia umana

valutato anche dopo aver ascoltato le parole del Governo che - sono convinto - in tempi rapidissimi vorrà essere presente in Aula per fornire elementi di dettaglio in merito a quello che è troppo semplice

Il nostro Paese è sicuramente tra quelli più performanti, in Europa, per quanto riguarda l'alta velocità;

Dovremmo impegnare la politica in maniera giudiziosa affinché non si arrivi, come oggi, a contare decine di vittime. Speriamo che il conto si fermi alle 20 vittime riportate

Signor Presidente, questo è il momento del cordoglio e noi siamo vicini alle famiglie delle vittime a quanti stanno tribolando per la sorte dei feriti. Diciamo un grazie sentito a quanti sul posto stanno svolgendo il loro lavoro, come servitori dello Stato o come volontari.

ha colto nei volti degli abitanti di quella Provincia e di quei Comuni, volti scavati come gli alberi degli ulivi che puntellano quel paesaggio e che riportano un vissuto che si rifà ad una civiltà contadina il cui tratto non è mai venuto meno e che la modernità non è mai riuscita ad eliminare. Viene in mente, vedendo le scene che abbiamo visto in televisione, di citare Tommaso Fiore e il suo popolo di formiche, quel popolo di persone laboriose, quel popolo di persone mai dome e mai stanche, quel popolo che può essere schiacciato da qualcosa di più grande che lo sovrasta. che lo sovrasta. Ecco, quel qualcosa di più grande lo possiamo rappresentare con l'antitesi tra il binario unico su cui viaggiavano i due treni e il *computer* che non ha funzionato. Qualcosa che ci riporta all'arretratezza di quelle terre e qualcosa di incredibilmente moderno. contrapposizione, signor Presidente, è il segno distintivo della Regione che forse più di ogni altra amo ed è il segno distintivo di tutto il Mezzogiorno. Ripeto che non è il momento della polemica e quindi queste parole non vogliono nemmeno in maniera velata richiamarla, ma di binario unico e della necessità di superarlo, noi che veniamo di lì abbiamo sentito parlare tutta la vita, da quando eravamo bambini ed è ancora oggi una tragica realtà. Credo, signor Presidente, che, se questa tragedia ha un senso, è anche quello di richiamare la nostra attenzione su una parte d'Italia, il Sud, che non può diventare quello che la Corsica è per la Francia: una palla al piede senza possibilità di riscatto. Il divario che cresce tra le diverse parti del Paese, invece, questo fa immaginare. Ma, se non cresce il Sud, non cresce l'Italia. Per questo, signor Presidente, questa è una tragedia che ancor di più colpisce tutto il Paese, le sue contraddizioni e i suoi ritardi. Chiedo infine, rinnovando i nostri sentimenti di cordoglio e di vicinanza,

Non è giusto dover dire addio a un figlio, a un padre, a una madre, a un amico. Non è tollerabile assistere inermi a una tragedia di queste dimensioni, che oggi ha scosso la mia Puglia, ha scosso l'Italia Non è possibile, no, non è possibile neppure che nei prossimi giorni, settimane e mesi si debba assistere al solito scaricabarile sulle responsabilità che, nella mattinata di oggi, hanno causato una delle più gravi tragedie vissute dalla mia Puglia in tempi moderni. È giusto che ora si pensi ai feriti, che si pensi alle vittime; sarà giusto nel prossimo immediato futuro garantire a chi soffre adeguata assistenza; sarà giusto altresì garantire tempi certi, responsabilità chiare: nomi e cognomi. Sarà necessario capire cosa è accaduto e promettere - questo è un impegno che lancio a tutte le istituzioni, al Governo, alla classe politica tutta - che quanto accaduto oggi non accadrà più. Ai feriti va il mio abbraccio, il mio e quello di tutta l'Assemblea del Senato, sia pure oggi un po' distratta e chiassosa, in un momento così difficile per tante famiglie e per l'Italia intera. Alle famiglie delle vittime va il nostro più sentito cordoglio e l'impegno a non lasciare impunita questa tragedia.

di fronte a tragedie di questo genere la semplice partecipazione e espressione di cordoglio per le vittime e verso le loro famiglie mi paiono assolutamente insufficienti e inadeguate. Il Parlamento e coloro che portano la responsabilità delle politiche generali del Paese non possono cavarsela, anche di fronte all'errore umano o a un guasto tecnologico, solo con il cordoglio

Credo che dovremmo riflettere su un punto: in un Paese moderno e avanzato come il nostro, di fronte a una tecnologia che consente di mettere in campo sistemi di sicurezza che garantiscono, se non il 100 per cento, il 99 per cento di quanto è necessario per dare agibilità sicura ai mezzi di trasporto, in particolare quelli ferroviari, come è possibile che su tratte sia pure non di primaria importanza, ma comunque importanti e che interessano migliaia di cittadini tutti i giorni, possano accadere vicende e fatti di questo genere? Credo dovremmo riflettere sulla necessità di orientare una maggiore attenzione sulle caratteristiche delle aziende che svolgono questa funzione, che sono aziende di carattere locale, sul fatto che molto spesso le professionalità messe in campo sono inadeguate o molto improvvisate, e anche sui carichi di lavoro, che probabilmente possono anche essere elevati in situazioni al limite, che spesso

possono essere doppi, si può arrivare a particolari raffinatezze e si può fare in modo che l'errore umano sia ridotto ai minimi termini. Voglio esprimere il cordoglio per questa tragedia, che si aggiunge ad altre tragedie a cui in questi giorni abbiamo dovuto assistere, ma che non dipendevano da noi perché sono accadute in altre parti del mondo e probabilmente sono state frutto di iniziative di soggetti

non deve essere vista come una speculazione del momento, bensì come una necessità di risoluzione del problema per il futuro. Presidente, non sappiamo ancora tutto sulle dimensioni del disastro disastro che si è verificato questa mattina nel tratto ferroviario tra Andria e Corato. Sappiamo, comunque, che tante sono le vittime finora accertate (forse 20, forse più) e tanti i feriti, che raccontano di una tragedia umana terribile e intollerabile. È per questo

il dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. Vogliamo ringraziare tutti coloro che operano nei soccorsi e che sono intervenuti, con grande tempestività, evitando che il conto di questo disastro fosse ancora più tragico. Ma se è vero, come pare, che quella tratta ferroviaria è stata interessata negli ultimi quindici anni da 120 incidenti, e che sono 70 le vittime e moltissimi i feriti che hanno accompagnato l'esistenza di quel segmento di ferrovia, penso che dobbiamo porci seriamente il problema e non liquidare le cause di questo incidente come riconducibili a un possibile errore umano. Evidentemente, le caratteristiche di quel tratto ferroviario sono tali da rendere insicuro

Tanti studenti, tanti lavoratori, tanti pendolari; i viaggiatori che utilizzano prevalentemente quel tratto di ferrovia (70 chilometri su un binario unico) raccontano, come è stato detto, di una condizione delle ferrovie, soprattutto delle ferrovie regionali, delle ferrovie locali, del trasporto pubblico locale del Mezzogiorno, ormai

di quelle terre e un disagio aggiuntivo per quelle popolazioni, ma costituisce un significativo elemento di rischio, che mette in pericolo la vita di coloro che operano operano in quel servizio e di coloro che quel servizio utilizzano. Vorremmo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, appena possibile, il ministro Delrio venisse in Parlamento, in quest'Aula, a riferire in maniera esaustiva sulla tragedia, sulle sue proporzioni, ma anche sulle sue ragioni: su quelle immediate e su quelle antiche. Ecco perché, riproponendo la vicinanza più sincera alle famiglie delle vittime e ai feriti, noi, signor Presidente, chiediamo che il Governo, nel più breve tempo possibile, si presenti in Senato.

dell'augurio a tutti i feriti di potere ristabilirsi al più presto e della fraterna solidarietà a tutti coloro che nel gravissimo incidente sono sopravvissuti.

contenere, nei limiti del possibile, i danni già enormemente gravi di questo incidente. Questo è il sentimento che prevale in chi, come me, conosce molto bene quella linea, perché attraversa praticamente tutti i paesi limitrofi al mio

Conosco quanto a rilento siano andati i lavori in un primo tratto e presso le stazioni di un secondo binario e so perfettamente che quella parte è ancora a binario unico. il dolore, l'auspicio per il ristabilimento dei feriti, il cordoglio per i familiari e la solidarietà per i sopravvissuti, adesso bisognerà occuparsi presto della questione. Le responsabilità andranno accertate con rapidità dagli organi competenti e i provvedimenti conseguenti andranno presi con altrettanta rapidità, ma noi, uomini della politica e delle istituzioni,

Lo dico così, perché conosco quella linea: ci sono ancora decine di passaggi a livello praticamente incustoditi e tutti attraversano così quella linea.

per onorare tutti coloro che, purtroppo, sono deceduti o che in questo momento sono feriti, è quello di fare in modo che questo non accada più e questo sarà il nostro compito.

e che, soprattutto, nessun orpello burocratico sia frapposto ad un rapido incedere dei lavori. Spero che il

ci associamo ovviamente al cordoglio. Non ci sono parole per esprimere quello che è accaduto questa mattina e per descrivere questa tragedia. Ovviamente il nostro primo pensiero va alle vittime e alle famiglie delle vittime. Parliamo di più di venti morti e più di trenta feriti. È in questo momento che occorre chiedere al Governo, in particolare, di assicurare e di svolgere qualsiasi attività per dimostrare vicinanza e conforto, anche materiale, alle famiglie. Un ringraziamento doveroso va ai sanitari che in questo momento stanno prestando i soccorsi ai feriti e ai donatori pugliesi che si stanno recando ad effettuare donazioni di sangue per l'emergenza che si è creata. Nel 2016 accade accade che su un solo binario due treni a più di cento chilometri all'ora si scontrino: questo non può accadere. Oggi il cordoglio non può più bastare. Questa è l'ennesima tragedia, signor Presidente, che ha colpito il Mezzogiorno d'Italia. La nostra, la mia amata Puglia, protagonista di un vergognoso caso di inefficienza e di insicurezza del sistema del trasporto pubblico locale. Mentre al Nord si sperperano soldi per la TAV, il Sud è costretto a convivere ancora con reti ferroviarie affidate a strumenti di sicurezza ormai superati, con binari unici,

l'alternanza tra treni provenienti da direttrici opposte fosse regolata attraverso comunicazioni telefoniche: uno scandalo. Oggi siamo qui a piangere la morte ingiusta dei nostri cittadini che hanno avuto fiducia nello Stato. Dobbiamo riflettere sulle priorità vere della nostra Italia, in particolare del Mezzogiorno: non è possibile che i nostri ragazzi, pendolari, lavoratori debbano vivere in luoghi così insicuri e inefficienti. Prima di scardinare le nostre montagne per opere superflue, pensiamo a garantire i servizi essenziali per i nostri cittadini: è un nostro dovere, è il dovere di una classe politica verso persone che non meritano di perdere la vita per l'inefficienza dello Stato e delle Regioni. È ora di finirla con questa vergogna: l'Italia e gli italiani meritano altro.

Vorrei anch'io esprimere in quest'Aula i miei sentimenti di vicinanza e di solidarietà alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia, che da pugliese mi tocca molto da vicino. Sappiamo che i soccorritori stanno operando in condizioni difficili e li esortiamo a fare tutto il possibile per salvare i feriti. Venti è il numero attuale delle vittime, ma da notizie certe che mi arrivano il numero purtroppo è destinato a salire. Le immagini dello scontro che abbiamo potuto vedere sono devastanti e ci lasciano senza parole. Conosco la sensibilità del ministro Delrio e sono certo, quindi, che si adopererà con la massima celerità e il per accertare i fatti fino in fondo e per aumentare la sicurezza del trasporto ferroviario nella mia Regione, perché ciò che è avvenuto lascia davvero sgomenti. Una domanda mi pongo: due treni sullo stesso binario che corrono l'uno contro l'altro. Com'è è stato possibile? E la burocrazia da anni ferma l'elettrificazione e il telecontrollo di quella tratta. Non è possibile. Oggi è il momento del silenzio e delle preghiere, della solidarietà e della vicinanza ai feriti e ai familiari, che non possono essere lasciati soli. Ho sentito i colleghi che sono intervenuti prima di me, senatori di altri partiti, ma oggi dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, dalla parte di chi ha preso un treno - che, vi assicuro, prendo anche io - per andare al lavoro, a studiare o magari in vacanza e purtroppo ha trovato la morte. Ringrazio per aver voluto cominciare la seduta odierna proprio con la sciagura ferroviaria avvenuta in Puglia ed esorto lei, Presidente, e tutti i colleghi a fare in modo che questa commemorazione non sia fine a se stessa,

Ripeto: non possiamo lasciarli soli, perché troppe volte al fragore della tragedia è seguito il silenzio dell'abbandono. Spente le telecamere, purtroppo tutto è stato dimenticato. Se la politica ha un senso, è proprio quello di essere vicina alle persone in difficoltà. Dobbiamo capire quello che è successo perché incidenti del genere non abbiano più a verificarsi, ma questo lo faremo domani. Oggi piangiamo le vittime innocenti, alle cui famiglie rinnovo la mia vicinanza e quella di tutto il Gruppo di Forza Italia.

il più vivo cordoglio per le vittime dell'immane tragedia che si è consumata nelle scorse ore in Puglia tra le città di Andria e Corato, dove - come hanno ricordato numerosi colleghi - a seguito dello scontro frontale tra due treni delle Ferrovie del Nord Barese, hanno perso la vita al momento oltre 20 persone e numerosi sono i feriti, tra cui alcuni gravi. In questi istanti il nostro primo triste pensiero va a loro, alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti, in quello che appare ancora un bilancio tragicamente provvisorio

tra le lamiere divelte dei convogli distrutti da un impatto così violento, e abbiamo dinanzi a noi l'immagine di quel bambino salvato da questo così tragico incidente.

di salute, di spesa o per ricongiungersi con i propri familiari, presso il capoluogo pugliese. Si tratta di un gravissimo incidente le cui cause al momento pare siano ancora in gran parte inspiegabili:

il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Graziano Delrio, per coordinare i soccorsi e avviare le necessarie attività di indagine, che credo i tecnici delle varie autorità

meritano con urgenza e che, siamo certi, appena possibile, il Governo verrà a riferire in queste Aule parlamentari. Il nostro auspicio e il nostro pressante invito al Governo e alle istituzioni coinvolte è che venga fatta chiarezza quanto prima e che vengano accertate tutte le responsabilità del caso. Ci conforta in questo senso la perentorietà con cui il Presidente del Consiglio nelle scorse ore, prima di recarsi sul luogo di questo così grave incidente, ha assunto l'impegno a favorire l'accertamento delle responsabilità. Verrà il tempo colleghi per interrogarci sull'adeguatezza della rete ferroviaria italiana in alcuni tratti della nostra penisola e di come è possibile che ancora oggi, con tutte le tecnologie disponibili, possano accadere questo tipo di tragedie, e nessun dubbio potrà essere evaso di fronte a ciò che è accaduto. Verrà il tempo perché tutti insieme si assuma come obiettivo prioritario quello della qualificazione, del potenziamento e dell'ammodernamento delle reti e delle linee che quotidianamente milioni di italiani utilizzano da pendolari, al pari dello sforzo straordinario che in questi ultimi decenni il Paese ha compiuto attorno all'Alta velocità. Verrà questo tempo. Nel frattempo, in questi minuti, in queste ore, è il tempo per tutti noi di raccogliere le nostre forze in un sentimento di dolore e cordoglio per le vittime, di solidarietà alle loro famiglie, di apprensione e di vicinanza ai tanti feriti.

riferito in Commissione che avremmo cercato di acclarare quello che era accaduto, naturalmente anche per poterne parlare con i colleghi della Commissione stessa. Naturalmente anch'io esprimo profondo cordoglio nei confronti delle famiglie che sono state così pesantemente colpite. Non siamo abituati per nostra cultura, quando avviene una tragedia così immane, ad individuare immediatamente chi sono i colpevoli, ma siamo più portati a pensare come assistere e cercare di trovare una soluzione che possa possa salvare più vite umane possibili. Certo - lo hanno ripetuto già altri colleghi - è un fatto incredibile come con le nuove tecnologie non si possano individuare due treni che vanno sulla stessa linea uno contro l'altro. Ma questo lo acclareremo nei prossimi giorni. Ho apprezzato molto il fatto che il ministro Delrio si sia immediatamente recato sul posto, perché così deve fare un Governo e di questo ne voglio dare atto. Sicuramente, vista la sua sensibilità, verrà a riferire in Parlamento e spero che voglia riferire anche nell'ambito della Commissione, perché dovremmo cercare di trovare alcune soluzioni. Noi abbiamo una linea ferroviaria

che RFI gestisce su tutto il territorio nazionale. Qualche controllo in più dobbiamo sicuramente disporlo, tutti insieme, e non è necessario

Mi associo inoltre alle sue dichiarazioni, Presidente, e a nome del Presidente del Consiglio e dell'interno Governo esprimo grande cordoglio per le vittime, solidarietà alle famiglie e grande vicinanza ai numerosi feriti. L'incidente è per caratteristiche e proporzioni di considerevole impatto. Le cause sono in via di accertamento, come i colleghi hanno detto; penso che ogni conclusione ora, allo stato dell'arte, sia assolutamente impropria. I tecnici del Ministero e della società ferroviaria sono già sul posto per comprendere le dinamiche e, come è stato detto poc'anzi, il ministro Delrio è sul posto per

assai probabilmente già nella giornata di domani, previa intesa con la Presidenza del Senato. ringraziare in modo particolare i soccorritori che si stanno prodigando in queste ore, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, gli assistenti sanitari, i volontari, la Protezione civile e i donatori di sangue che sono, come sempre, espressione dell'Italia migliore. ci saranno elementi utili per riprendere questa dolorosa, ma doverosa discussione. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato - salvo questa vicenda che affronteremo sicuramente - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 agosto. Nella seduta di oggi inizierà la discussione del disegno di legge sulla modifica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Per tale provvedimento è previsto il voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Le dichiarazioni di voto avranno luogo domani, alle ore 16,30. Pertanto, la Presidenza è stata autorizzata all'armonizzazione dei tempi. Su richiesta di due Gruppi parlamentari, la seduta unica di domani sarà sospesa alle ore 12 e riprenderà alle ore 15, senza orario di chiusura, al fine di consentire la votazione a scrutinio segreto delle dimissioni presentate dal senatore Vacciano e l'esame del disegno di legge in quarta lettura in materia di missioni internazionali. Giovedì proseguirà l'esame del disegno di legge sul delitto di tortura e seguiranno poi gli argomenti già previsti dal calendario vigente, anticipando il disegno di legge

su organizzazione degli uffici giudiziari e situazione del personale amministrativo, nonché sulle condizioni delle carceri. Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni, nonché con l'esame del rendiconto e del bilancio interno del Senato. Fermi restando gli altri argomenti già previsti, il calendario della settimana dal 26 al 28 luglio è integrato con 1'esame del disegno di legge di riforma del processo penale, nonché con due decreti-legge presentati alla Camera dei deputati in materia di finanza degli enti locali e processo amministrativo telematico.

Signor Presidente, noi non siamo assolutamente d'accordo, come abbiamo già evidenziato nella riunione dei Capigruppo, sull'inversione che si è prodotta, ed è stata

sulla tortura che, vorrei ricordare, è stato sepolto in Commissione giustizia per molto tempo,

alla modifica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, francamente a noi è sembrato non tanto finalizzato ad approvare rapidamente questo disegno di legge, legge, previsto comunque per domani, ma, ancora una volta, un tentativo - ci dispiace dirlo - di far naufragare l'approvazione del disegno di legge sul delitto di tortura. Vorrei ricordare a tutti quanti che siamo in un ritardo spaventoso.

del documento XXII n. 33 per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul caso Regeni.

*(M5S)*. Signor Presidente, confermo quanto già detto nella Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo contestato la richiesta di inversione del calendario per due motivi fondamentali. Innanzi tutto vogliamo segnalare il fatto che il posticipo richiesto sulla discussione e sulla votazione del disegno di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento è semplicemente dettato da un problema che ha la maggioranza di discussione

quindi di proseguire con la discussione sul delitto di tortura. Abbiamo anche contestato questa inversione per un altro motivo e cioè che la maggioranza qualificata richiesta per il prossimo provvedimento, in realtà, riuscite a garantirla soltanto il mercoledì

vostri elementi e non squalificata da altri che vi vengono in soccorso. Questa è una dura critica che vi faccio. Siete in grado di mantenere la maggioranza qualificata soltanto il mercoledì e non avete il coraggio di assumervi le vostre responsabilità rigettando quella che magari ritenete una maggioranza squalificata. Visto che il calendario

Comunico all'Assemblea che, con tre distinte lettere, il senatore Luis Alberto Orellana ha chiesto di promuovere, ai sensi dell'articolo 6

«Approvate voi il testo, diviso per parti separate e omogenee, della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento dei bicameralismo paritario, la riduzione dei numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,

nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 88 dei 15 aprile 2016, 2) «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 88 del 15 aprile 2016, nella parte in cui, all'articolo 15, modifica l'articolo 75 della Costituzione relativo al *referendum* abrogativo?». «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione dei CNEL e la revisione dei Titolo V della parte II della Costituzione",

commi da 1 a 6, modifica l'articolo 57 della Costituzione, relativo alla composizione e all'elezione del Senato, e le disposizioni connesse?». In tutte e tre le lettere sono indicati, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, quali delegati a depositare le richieste di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione i senatori Lorenzo Battista, Serenella Fucksia e Luis Alberto Orellana. Il *quorum* per la presentazione delle richieste di *referendum* è di 65 firme. Le richieste dovranno pervenire alla Cancelleria della Corte di cassazione entro il 15 aprile 2016. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i senatori che intendano sottoscrivere le suddette richieste di *referendum* potranno recarsi presso il Servizio dell'Assemblea del Senato a partire dalle ore 18 di oggi fino alle ore 20,30. Da domani le richieste potranno essere sottoscritte dalle ore 9,30 alle ore 20. I funzionari delegati dal Segretario Generale provvederanno all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori.

Presidente, volevo segnalare che, nel dare lettura della possibilità di firmare per il *referendum*, lei ha indicato come data di scadenza, per errore materiale, il 15 aprile. In effetti, la data è il 15 luglio, cioè venerdì prossimo. Altra considerazione che volevo fare è la

alla cancelleria della Corte di cassazione entro il 15 luglio. Probabilmente, si fa confusione con il fatto che il 15 aprile è stato il giorno di pubblicazione

Signor Presidente, senatrici, senatori, il disegno di legge "enti locali", come da molti è sinteticamente chiamato, prevede modifiche alla legge n. attuativa del principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione. Ricordo però che tale legge fu emanata in un contesto storico, politico e congiunturale molto diverso dall'attuale, anche se sono passati pochi anni. L'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede il vincolo dell'equilibrio di bilancio, non deve diventare però un vincolo amministrativo burocratico eccessivo e, soprattutto, non deve diventare un impedimento per le autonomie locali, nella loro discrezionalità e capacità programmatoria, soprattutto per quanto attiene agli investimenti. L'importante ruolo di motore di sviluppo e investimenti su tutto il territorio nazionale degli enti locali non va mortificato, soprattutto in questi anni in cui il massimo impegno va rivolto alla crescita e al superamento della crisi. Si tratta di modifiche, per così dire, "di sistema". In primo luogo c'è il definitivo superamento del Patto di stabilità. Sono modifiche strutturali, che ritengo molto importanti e che devono trovare la più ampia condivisione, perché andranno applicate e sostenute indipendentemente dalla maggioranza di Governo e in tale direzione ho svolto il mio ruolo di relatrice. Il disegno di legge prevede innovazioni importanti, molto attese dagli enti territoriali. propone di semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento, raccordando le norme approvate in questi anni; di semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibrio di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali, consentendo altresì una politica espansiva. semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, dall'altro, le modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo sempre conto della recente sentenza della Corte costituzionale. In un'unica parola, il messaggio più grande è: semplificare la vita agli enti locali e soprattutto consentire investimenti. Per quanto riguarda il contenuto preciso dei quattro articoli, rinvio alla relazione illustrativa stampata nel fascicolo dell'Assemblea, per non appesantire la serata. Ricordo solo sinteticamente che l'articolo 1 sostituisce i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle Regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Questo significa ridurre fortemente i vincoli. L'articolo 2, prevede modifiche alle norme, per lo più procedurali, che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Gli articoli 3 e 4, infine, semplificano le disposizioni vigenti in tema di concorso degli enti territoriali al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, nonché in tema di concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico. Sembrano parole complicate, ma in realtà significano davvero semplificazioni per i Comuni e gli enti territoriali. L'importanza delle innovazioni e delle semplificazioni contenute nel disegno di legge è stata apprezzata sia dai soggetti auditi che dai Gruppi di maggioranza e di opposizione. Come sempre, però, ogni provvedimento può essere migliorato in sede parlamentare. A seguito delle audizioni, avvenute congiuntamente tra Camera e Senato, è stato presentato un numero contenuto di emendamenti, che denota anche la volontà non ostruzionistica delle opposizioni riferimento ad alcuni temi sottolineati dagli enti territoriali auditi; emendamenti che sono stati presentati identici o simili da quasi tutti i Gruppi parlamentari. Il lavoro in Commissione, con l'apporto dei Gruppi di maggioranza, dei Gruppi di opposizione e del Governo, ha portato alla stesura di due emendamenti da parte della relatrice che sono stati approvati all'unanimità, e voglio sottolinearlo; infatti, quando si parla di enti territoriali la sensibilità è trasversale e la ricerca delle migliori soluzioni ci trova sempre disponibili a raggiungere un accordo. Purtroppo alcune istanze (ad esempio quelle sull'utilizzo dell'avanzo), pur fortemente condivise dalla sottoscritta, non hanno potuto essere accolte perché richiedevano una copertura finanziaria impossibile da trovare allo stato attuale oppure perché inammissibili per materia. Ma sono fiduciosa che potranno essere accolte, in tutto o in parte, nei prossimi provvedimenti. Gli emendamenti approvati all'unanimità riguardano una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale vincolato negli anni 2017-2019 sarà introdotto fra le entrate e le spese spese finali secondo quanto stabilito con la prossima legge triennale di bilancio. La fase transitoria risulta indispensabile in quanto i fondi pluriennali vincolati degli enti territoriali sono corposi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e la loro applicazione necessita di una graduale inserimento sul lato delle entrate. Al termine del bilancio triennale 2017-2019 si entrerà in una fase a regime in cui il fondo pluriennale vincolato è introdotto in via permanente fra le entrate finali e le spese finali degli enti territoriali. Questo vuol dire moltissimo per gli enti territoriali: significa la possibilità di fare investimenti. Gli investimenti a livello locale sono ripresi in quest'ultimo anno e questa è un'ulteriore boccata di ossigeno. Ci sarà poi un accordo tra l'ANCI e il Governo anche per quanto riguarda le cifre che potranno essere inserite nel prossimo bilancio, ma sicuramente aiuteranno ad aumentare gli investimenti. altro emendamento approvato all'unanimità trae origine dalla riformulazione di un emendamento richiesto dalla Commissione, con il quale si prevede che le operazioni di indebitamento e d'investimento, realizzate dagli enti locali attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e non soddisfatti dalle intese regionali, sono effettuate sulla base di appositi patti di solidarietà nazionali. La norma introduce un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, facendo ovviamente salvi gli effetti di tale strumento nazionale rispetto all'invarianza del fondo finale del complesso degli enti territoriali. Anche questo, in estrema sintesi e semplificazione, vuol dire liberare risorse per gli enti locali e di nuovo in particolare sugli investimenti.

come la legge di stabilità 2016 e i decreti-legge enti locali (quello dell'anno scorso e quello in questo momento all'esame della Camera), che stanno progressivamente delineando un percorso di normalizzazione dell'attività degli enti territoriali. Stiamo quindi tornando gradualmente a un regime di normalità, almeno nelle procedure: la conoscenza delle regole per la stesura dei bilanci di previsione ne consente la loro approvazione nei tempi corretti, ovvero entro dicembre o al massimo febbraio, rientrando progressivamente dalle scadenze anomale che abbiamo visto nel triennio 2013-2015, in cui si era arrivati addirittura ad approvare i bilanci entro novembre dell'anno in corso.

e il Governo, per la disponibilità a modificare il testo iniziale e per il contributo fornito nella ricerca delle soluzioni tecniche possibili.

Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge reca una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 (Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico), dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare ai sensi della citata legge con il nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali. Ebbene, in altri tempi con un titolo del genere il disegno di legge avrebbe annunciato l'ennesima stangata per gli enti locali; una serie di regole meccanismi burocratico-contabili tesi a imbrigliarne le capacità e le possibilità di programmazione, a limitarne la spesa e, soprattutto, nell'ultimo periodo, anche a residuare un avanzo destinato all'abbattimento dei debiti. Oggi il provvedimento ha un segno e un colore decisamente opposti. Con questo provvedimento si pone fine semmai alla lunga stagione nel corso della quale concordemente con le amministrazioni centrali, hanno dovuto contribuire - e con un prezzo pesante - al risanamento dei conti pubblici attraverso i meccanismi del Patto di stabilità interno. Enti locali che spesso sono stati sacrificati in questo rapporto con lo Stato centrale e ciò ha determinato sostanzialmente sui territori l'impossibilità di programmazione e il drastico calo, per non dire

questo provvedimento, che si accompagna all'ultima legge di stabilità, pone fine in maniera definitiva - sebbene con una

piena capacità programmatoria e libera soldi per gli investimenti. Quindi, è una buona notizia per le amministrazioni locali e per l'economia, perché sappiamo che la ripresa degli investimenti pubblici concorre in maniera fondamentale alla ripresa del PIL nazionale. A queste misure largamente di segno positivo inoltre si aggiunge, attraverso il rafforzamento dei patti regionalizzati, l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio, sia attraverso il ricorso al debito mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, sia rafforzando il ruolo Chiudiamo un'epoca e lo facciamo sommessamente, mentre per molti anni, in maniera molto meno sommessa, si è inveito

questo traguardo storico, che fino all'anno scorso era impensabile e non annunciato. Tuttavia non ci illudiamo, ma quantomeno ci auguriamo che il Parlamento sottolinei

Poniamo fine alla gestione dei farraginosi saldi: i quattro saldi di riferimento dei bilanci di Regioni e enti locali sono sostituiti da un unico saldo, non negativo, ma solo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono conseguentemente soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti: questo significa semplificazione. Ma soprattutto - questo ha invece un valore sostanziale ben più importante - con la lettera *b)* si dispone l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato: un fondo importante a cui i nostri amministratori si abitueranno ben volentieri, perché significa superamento dei limiti precedenti del Patto di stabilità. Questo fondo, che riguarda l'entrata e la spesa, è un saldo finanziario costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive (tipicamente le opere pubbliche dell'ente già impegnate) ma esigibili esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo, dal punto di vista contabile, ha l'obiettivo di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. In altre parole, l'effetto che tutti avevano imparato a conoscere per cui viene contratto un mutuo ma le spese vengono sostenute negli anni successivi creando uno squilibrio è, dal punto di vista contabile, rimediato pienamente dal fondo. Le risorse del fondo pluriennale però sono destinate destinate prevalentemente alla spesa in conto capitale, ma anche per la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Il fondo pluriennale risulta immediatamente immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano. È possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo. In questo modo si liberano risorse e si può tornare a fare una sana programmazione. Segnalo, infine, che l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell'equilibrio complessivo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando, come anticipato, una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. l'eventuale rientro nel caso in cui un ente territoriale registri un valore negativo del saldo. Il rientro precedentemente era previsto in tre anni senza alcun tipo di vincolo. Ci è parso opportuno, in questa sede, precisare che nel triennio successivo si debba rientrare in quote costanti. Naturalmente il motivo è abbastanza evidente: si è di fronte al tradizionale *trade off* tra lasciare completa libertà alle amministrazioni locali senza dare alcun principio e, quindi, lasciare alla responsabilità dei singoli amministratori anche le scelte puntuali oppure introdurre principi di buonsenso, tesi a evitare squilibri tra le annualità, particolarmente anticipatici e fastidiosi, allorquando, in questo periodo, ci fosse un cambio di amministrazione. In altre parole, in questo caso la scelta è di di imporre un'equità nell'ambito del triennio piuttosto che assistere allo scaricabarile sul futuro. Forse, in questo caso, lo Stato dimostra buonsenso più che un'imposizione di termini. Signora Presidente, credo che sia giusto sottolineare come questo provvedimento come questo provvedimento segni la fine di un periodo di forte difficoltà nell'amministrazione finanziaria degli enti locali, riconsegni la capacità di programmazione e incida anche sulla possibilità di ripresa del nostro Paese. Colleghe e colleghi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti renderà un'informativa al Senato sul grave incidente ferroviario accaduto domani, alle ore 18,30, dopo il voto finale sul disegno di legge in materia di bilanci degli enti locali.

Signora Presidente, il presente provvedimento modifica la legge sul pareggio di bilancio degli enti territoriali. territoriali. Come ha detto la relatrice, è certamente un provvedimento atteso quanto innovativo che consente una semplificazione rilevante della contabilità pubblica. Rende maggiormente gestibile il passaggio dal Patto di stabilità al pareggio di bilancio ed elimina alcuni vincoli che rendevano più rigida e complicata la programmazione della spesa e degli investimenti. Ora, si tratta di un provvedimento di adeguamento tecnico, questo è evidente, che però ha un elevato valore politico

comprese le Regioni, mediante l'attribuzione di elementi di finanza pubblica coerenti con il nuovo ordinamento contabile, una gestione più efficace delle risorse, tenendo conto delle specificità di ogni ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. attraverso un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge cerca di raggiungere l'obiettivo di favorire l'aumento degli investimenti sul territorio, come avevano detto già altri colleghi, sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e, in qualche modo, anche attraverso il ruolo delle Regioni come cabine di regia nell'ambito del proprio territorio di riferimento. In sostanza, alla fine il testo semplifica complessivamente il quadro normativo in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e ridefinisce anche come questi concorrano alla sostenibilità del debito pubblico. Le modifiche contenute in questo disegno di legge si articolano su alcune direttrici di intervento. Mi concentrerò soprattutto sulla prima, che riguarda l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali.

siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Quindi, sono soppressi tutti gli obblighi di pareggio di cassa e quello delle spese correnti. Questo semplifica molto la vita degli enti locali e la semplifica perché è complesso, in fase di passaggio, pensare di avere pronti i quattro saldi di riferimento e soprattutto

con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa tra le entrate finali e le spese finali. abbiamo finalmente uno strumento di indubbia efficacia e competitività che consente di rilanciare gli investimenti da parte dei Comuni e delle Regioni, eliminando definitivamente quella gestione distorta che si è formata nel tempo con i residui attivi e passivi che

alle Regioni che avevano avviato già il pareggio di bilancio in anticipo si era chiesto di pensare ad una forma di flessibilità per l'utilizzo nel triennio di tali risorse. Il Governo, tuttavia, non aveva trovato le risorse per poterlo fare, anche perché si trattava di un elemento incentrato sulle Regioni che sperimentalmente, parlo di alcune

ai bilanci di previsione, tuttavia va detto che in questo momento, alle condizioni date, questo è certamente un passo in avanti importante per tutti i Comuni. Le risorse del fondo fondo sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma attraverso la norma in esame si può andare anche a garantire la copertura delle spese correnti pur con alcuni vincoli. Il fondo triennale ha il vantaggio di essere immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili già nell'esercizio in corso e anche negli esercizi successivi. con questo fondo abbiamo finalmente uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo. citare alcuni elementi di maggiore flessibilità che riguardano il recupero flessibile non in quote costanti di un valore negativo del saldo, la soppressione del vincolo di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione di un debito maturato dall'ente al finanziamento in spese di investimento e, infine, il cambiamento del sistema sanzionatorio in un sistema che adesso non è più sanzionatorio in senso stretto, ma premiante per gli enti locali, stabilito con legge dello Stato che prevede che prevede non soltanto sanzioni, ma anche la possibilità di premiare gli enti locali virtuosi che mettono a disposizione una parte del margine di flessibilità.

incontro alle difficoltà dei Comuni più piccoli che non hanno risorse umani tali da poter dedicare tempo in eccesso alla complessità di operazioni che, invece, attraverso questo lavoro, vengono semplificate. In particolare

anche l'utilizzo dell'avanzo di esercizi precedenti per operazioni di investimento e, in questo senso, costituisce anch'essa un ulteriore elemento di flessibilità.

n. 243, intervenendo in tema di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Mi auguro, per la mia esperienza di amministratore locale ancor più che in qualità di senatore,

da fasi di sperimentazione e continue modifiche normative nell'ottica del superamento del Patto di stabilità interno. Di certo, una critica generale al disegno di legge in esame deve essermi consentita. Come la stessa Corte dei conti ha rilevato nel corso delle audizioni in Commissione bilancio, il presente disegno di legge, piuttosto che cercare di adattare i contenuti della riforma contabile dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011

della Costituzione, persegue il coordinamento tra le due normative, adeguando all'opposto i vincoli di finanza pubblica ai nuovi principi contabili. Ma vi è di più. L'idea dello Stato autosufficiente e sovrano è smentita dalla realtà dei fatti. Lo Stato, al pari di qualsiasi altro debitore, deve dimostrare di essere in grado di rimborsare il suo debito, soprattutto quando gli investitori sono in larga misura stranieri. E proprio la sottoposizione ad un sistema di relazioni internazionali, basata su una mutua accettazione di comportamenti nei mercati internazionali, ha determinato la necessità di introdurre meccanismi di limitazioni strutturali della spesa pubblica, in modo da consentire nel lungo periodo la sostenibilità e la rimborsabilità del debito. Per tali ragioni, gli Stati aderenti all'Unione europea hanno firmato nel 2011 un trattato internazionale noto ai più con il nome di *fiscal compact*, attuato in Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012, cui è seguita la già citata legge di attuazione n. La legge n. 243 introduce - come è noto - nella normativa italiana, in modo costituzionalmente "rafforzato", obblighi di pareggio di bilancio derivanti dalla situazione di gravissima instabilità della finanza pubblica che il Paese ha affrontato dalla fine del 2011. Le formulazioni allora adottate, con particolare riferimento agli enti territoriali, hanno delineato uno scenario eccessivamente restrittivo, marcatamente centralistico, finanche dell'autonomia di entrata e di spesa di cui i Comuni godono in forza del dettato costituzionale, ed incapace di incorporare le novità che di lì a poco sarebbero state introdotte dalla riforma della contabilità pubblica. Di certo è ad oggi opportuno modificare la legge n. 243, proprio per superare i limiti del disegno iniziale e per assicurare una maggiore flessibilità nella capacità di gestione dei contributi al risanamento e alla crescita. Allo stesso tempo, però, non si può non sottolineare che i continui mutamenti normativi riducono inevitabilmente la capacità programmatoria dei nostri Comuni, che al contrario dovrebbero essere posti in condizione di operare in un contesto di regole certe e stabili nel tempo. Per favore, riposizioniamo, dopo lustri di indifferenza, la nostra attenzione agli enti locali. Essi sono l'anima della nazione, il *front office* dello Stato nei confronti dei cittadini, ed incarnano l'idea tutta italiana della comunità. Dovremmo avere il coraggio di chiederci, e chiedo al Governo di fare altrettanto, se la colpa per l'assenza di programmazione sia dei burocrati, che si limitano ad attuare le disposizioni di legge, o non sia piuttosto del legislatore, che quelle regole continuamente continuamente muta. In questa sede voglio sottolineare un altro dato. Gli *slogan* governativi indicano proprio negli enti territoriali la fonte della spesa e degli sprechi pubblici. La prevista ed ancora non attuata abolizione delle Province sarebbe giustificata anche da tale esigenza. La realtà è ben altra. Secondo uno studio condotto nel giugno di quest'anno dal Centro studi e ricerche Unimpresa, il debito degli enti locali è diminuito del 14 per cento, mentre quello delle amministrazioni centrali è salito del 5 per cento. Per entrare nel dettaglio, da aprile 2014 a marzo 2016 il debito delle pubbliche amministrazioni territoriali è passato da 107 miliardi a 92 miliardi, con una riduzione generalizzata che ha interessato soprattutto i Comuni (che hanno ridotto il loro debito di ben 3 miliardi) rispetto alle Province (per le quali la riduzione del debito si è assestata a 643 milioni). All'inverso, il debito dello Stato è passato, nello stesso periodo, da 2.039 miliardi a 2.136 miliardi di euro. Secondo lo studio di Unimpresa, a pesare sul bilancio dello Stato sarebbero i costi dell'apparato statale, che rimangono in crescita permanente. Preso atto della realtà oggettiva, cui ho fatto breve cenno, vorrei ricordare a quest'Assemblea che il Gruppo Conservatori e Riformisti ha presentato tre emendamenti. Accolto con favore l'intento semplificatorio del disegno di legge in commento che sostituisce i vincoli di competenza e cassa attualmente previsti con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali e le spese finali, abbiamo proposto di inserire, a partire dal bilancio di esercizio del 2017, in modo strutturale, il fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati rilevanti ai fini tra gli aggregati rilevanti ai fini del nuovo saldo finale di competenza, soprattutto allo scopo di dare continuità al processo di rilancio degli investimenti locali faticosamente avviato con la legge di stabilità 2016. In secondo luogo, abbiamo proposto l'introduzione di uno strumento che consenta la redistribuzione dei vincoli di finanza pubblica su scala nazionale, prevedendo, altresì, un meccanismo di solidarietà nazionale che consenta il completo utilizzo delle risorse disponibili e riduca il rischio di vedere accentuate le distanze geografiche e dimensionali nell'ambito delle autonomie locali. In tal modo potrebbe realizzarsi una spinta agli investimenti locali senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. liberare risorse per gli investimenti, soprattutto in opere pubbliche, specialmente nel tribolato comparto delle infrastrutture, che, là dove realizzate, consentiranno di migliorare la mobilità e i collegamenti evitando - ad esempio che i treni continuino a viaggiare su un unico binario, come è accaduto questa mattina nella mia Puglia, causando l'immane tragedia

andiamo sostenendo da tempo: liberiamo risorse per garantire sicurezza ai cittadini, agli utenti, alle persone. il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà. legge n. 243 del 2012, che è legge rinforzata di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge n. 243, fatta dal Governo Monti alla fine del alla fine del 2012, aveva introdotto il principio del pareggio di bilancio per Regioni ed enti locali e il concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016. n. 243 aveva altresì introdotto l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri. Ricordo che, con la legge di stabilità 2015, il Governo Renzi aveva invece anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le Regioni a statuto ordinario, quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica in luogo del patto di stupidità, anzi del Patto di stabilità interno, incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali. Il provvedimento in esame è molto tecnico e vuole alleggerire i vincoli di bilancio degli enti territoriali modificando quattro articoli (dal 9 al 12) della legge n. 243, corrispondenti al Capo IV.

con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Vengono quindi soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti.

si prevede che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione. Vi sarà una intesa regionale anche per l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per le operazioni di investimento. L'articolo 3 modifica l'articolo 11 della legge n. 243 del 2012 (Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali). si demanda alla legge dello Stato il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Infine, c'è l'articolo 4, che modifica l'articolo 12 della legge n. 243 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico). Si tratta, dunque, norme positive, che introduce - come detto prima dalla relatrice Zanoni - modifiche di sistema, ma che poteva dare maggiori contributi positivi, come peraltro sottolineato

visti i molti mal di pancia all'interno della maggioranza traballante. La legge n. 243 può essere modificata, derogata o abrogata solo

Io non so se il provvedimento farà riprendere dall'agonia in cui sono precipitate Regioni, Province e Comuni, che da troppo tempo si trovano alle prese con una difficilissima e drammatica situazione finanziaria e organizzativa. Soprattutto dalla fine del 2011, grazie alle scelte operate dai Governi dei nominati Monti, Letta e Renzi con successive leggi di stabilità, vari provvedimenti legati all'emergenza e con operazioni elettorali di tipico stampo renziano, che irresponsabilmente hanno fatto schizzare alle stelle il debito pubblico,

Questo è, dunque, un provvedimento che tenta di riparare ai danni creati dall'Europa dei burocrati, concentrati a imporre solo stupida austerità con i parametri di Maastricht il *fiscal compact*, a cui - lo ricordo - solo la Lega Nord ha dato voto contrario; parametri che i Governi nostrani hanno subito, avallando e imponendoli al sistema delle autonomie locali.

di quasi il 40 per cento, contro il 13 per cento di riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali dello Stato. E tutte queste Regioni, ad eccezioni della Lombardia, hanno dovuto ricorrere all'aumento dell'addizionale regionale IRPEF. Stendiamo, poi, un velo pietoso sulle Province a seguito della demenziale riforma Delrio. In attesa dell'esito del *referendum* sulla riforma costituzionale, che Renzi e Boschi perderanno per l'arroganza e per il fallimento dell'azione di Governo, si registra un totale fallimento sulla semplificazione, visto che stanno nascendo modelli diversi in ogni Regione (vedi Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia). Si registra un marasma sul riordino delle funzioni e sul personale e, soprattutto, una vera emergenza sul lato delle risorse. Solo di tagli ai trasferimenti alle Province si è passati da 300 milioni di

Figuriamoci dunque come potranno affrontare le emergenze connesse al dissesto idrogeologico! Insomma, per le Province che vanno in dissesto regna il caos, perché è saltato completamente il legame tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzie di copertura finanziaria. Veniamo ora alle grida di dolore dei Comuni. In questi anni di risanamento dei conti della finanza pubblica i Comuni hanno fatto la parte del leone. Tra gli obiettivi del Patto di stabilità, i tagli ai trasferimenti e al fondo di solidarietà comunale, i Comuni hanno contribuito per 17 miliardi di euro, di cui solo 12,3 miliardi negli ultimi cinque anni.

È risultato inevitabile l'aumento della tassazione locale, con i sindaci chiamati a fare gli esattori per conto dello Stato. Sulla fiscalità degli immobili ricordo l'aumento da 9,2 miliardi di euro di gettito ICI del 2011 ai 25 miliardi di euro tra IMU e TASI del 2014, poi confermati nel 2015, di cui 4 miliardi di euro di gettito sugli immobili industriali, che - lo ricordo - andavano e vanno direttamente nelle casse ingorde dello Stato centrale. Caro *premier* Renzi, l'eliminazione quest'anno della TASI, introdotta e applicata da te e dal Partito Democratico, riporta il gettito sugli immobili a 21,5 miliardi di euro, ma il valore risulta ancora troppo alto. Siamo ormai al paradosso che diversi Comuni (molti di questi in Lombardia) non ricevono più i trasferimenti dallo Stato e vige una sorta di finanza decentrata al contrario, per cui le imposte locali riscosse dal sindaco vengono poi trasferite allo Stato. Mi avvio alle conclusioni: di questa grave situazione che tocca gli enti territoriali è doveroso sottolineare anche la conseguenza del calo drastico degli investimenti, con un taglio di oltre il 40 per cento, che per le Province. Si tratta di un'irresponsabile rinuncia a qualche punto di PIL e, dunque, una rinuncia a tante commesse di lavoro per le nostre imprese, sempre più stritolate dalla crisi economica e che continuano a morire, creando nuovi disoccupati, anche - e lo voglio ricordare - per eccesso di credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione, che è tutt'altro che azzerato, come invece aveva promesso Renzi

ed è risultata pressoché nulla la decantata lotta agli sprechi, di cui per molto tempo è andato blaterando Renzi, mentre si succedevano inefficaci commissari alla *spending review:* Cottarelli prima, Perotti poi e ora il consigliere economico Gutgeld.

ci si possa ritrovare in una situazione ulteriormente deteriorata: rischio, questo, molto alto con l'attuale Governo Renzi. È per tale ragione che questo Governo, con la sua compagine,

di legge provvede a modificare, in alcune sue parti, la legge n. 243 del 2012, cosiddetta "legge rinforzata", che reca «Disposizioni per l'attuazione dei principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione». In particolare, sono oggetto della proposta di modifica le disposizioni del Capo IV (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico). Il disegno di legge ha la finalità di adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso processi di semplificazione delle procedure. Nello specifico, ìl provvedimento sostituisce i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Inoltre, vengono disciplinate le operazioni di indebitamento e l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Infine, viene demandato a una legge statale il concorso delle autonomie alla sostenibilità del debito attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Ma facciamo ordine. legge n. 243 fu approvata, ai tempi del "Governissimo" Monti, da un Parlamento quasi coralmente prono all'Unione europea, che l'aveva imposta nel nome del rigore finanziario. Fra le richieste di Bruxelles, vi era anche quella di rafforzare i principi di sostenibilità dei bilanci pubblici, introducendoli nella Costituzione. A tal fine, venne varata la legge costituzionale n. 1 del 2012, di cui la legge n. 243 detta le disposizioni attuative. L'orrore del debito fu tradotto in una disciplina che non solo ha irrigidito la Costituzione, ma ha ridotto - oltre ogni ragionevolezza - i margini di manovra dei Governi, con l'evidente conseguenza di imporre politiche economiche ancora più restrittive. In particolare, ha messo seriamente in dubbio la possibilità di attuare le politiche sociali, che comunque trovano un riferimento nei nostri principi costituzionali. Hanno messo di fatto la Costituzione contro se stessa! L'iniziativa fu accompagnata da un clima punitivo, rovesciando sul cittadino le responsabilità di un intero ceto dirigente, imprenditoriale, politico e amministrativo. E le modifiche che si ispirarono alle dottrine dominanti della politica europea guidata dalla mannaia BCE ridussero al nulla assoluto le possibilità future di scelta delle politiche economiche e di progresso del nostro Paese. E infatti, il complesso dei vincoli imposti da questa disciplina si è rivelato una gabbia in grado di soffocare qualsiasi segnale di ripresa. In questo quadro, parrebbe inserirsi il disegno di legge licenziato dall'Esecutivo, che punterebbe ad alleggerire tale complesso di condizioni prima ancora che diventino vincolanti. La legge rinforzata n. 243 del 2012 costituisce l'attuazione della modifica costituzionale per l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, norma nei confronti della quale il Movimento 5 Stelle è sempre stato fortemente contrario. Pertanto, sebbene persista la nostra contrarietà verso l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, siamo tuttavia concordi nell'ammettere che esiste una necessità di riforma della legge Ma, nello stesso tempo, siamo convinti che in alcuni casi, come al solito, il rimedio che si intenderebbe porre ad alcune anomalie di questa legge è peggiore del male. Per tale motivo ci saremmo dovuti limitare a votare contro questo provvedimento. Tuttavia, abbiamo presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare alcune sue parti, soprattutto a favore della semplificazione delle regole di bilancio imposte per gli enti locali e dello stimolo agli investimenti da parte degli stessi. Particolarmente critiche appaiono - secondo noi - le modifiche recate dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Di fatto, le modifiche apportate agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 operano una semplificazione del meccanismo di perequazione civica previsto, eliminando ogni automatismo e sopprimendo l'obbligo sia di prevedere nel Documento di economia e finanza l'entità delle risorse da movimentare nelle diverse fasi del ciclo, sia di sottoporre al parere della Camera i criteri di riparto adottati. Non viene invece previsto, né nel testo vigente della citata legge n. 243 del 2012 né in quello risultante dalla revisione, che lo Stato debba trasferire alle amministrazioni locali una quota maggiore di capacità di spesa eventualmente derivante dall'applicazione delle clausole di flessibilità previste dalle regole europee,

definizione di una procedura celere flessibile per implementare gli investimenti. Occorre ricordare in ogni caso che il livello di finanziamento dello Stato ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché delle funzioni fondamentali, i cui *standard* sono definiti a livello centrale, deve essere calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, seppur definito da norme specifiche. I limiti della spesa pubblica sono stringenti e non si può non tenerne conto quando si definisce il livello delle prestazioni da erogare. Tuttavia, bisogna avere anche la consapevolezza che è impensabile definire i livelli essenziali di assistenza senza assicurarne contestualmente il finanziamento. In caso contrario, si farebbe ricadere la spesa solo su altri livelli di Governo, senza avere un beneficio a livello di finanza pubblica. La semplificazione procedurale proposta aumenta il margine di discrezionalità del Governo sulla misura dell'intervento per attenuare gli effetti del ciclo della finanza pubblica locale, cui fa fronte una maggiore incertezza sulle risorse a disposizione delle amministrazioni locali e, quindi, una riduzione della loro capacità di programmazione. Si deve, infine, rilevare come l'introduzione di numerosi rinvii alla legge ordinaria dello Stato, senza particolari delimitazioni degli ambiti di materia, non aiuti a disegnare quel quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi condivisi che la disciplina sull'equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe assicurare. La Costituzione, signora Presidente, è stata saggiamente prevista come un programma solidale: casa, lavoro, salute, istruzione, ambiente, giustizia. Tutto ha bisogno di interventi pubblici e poco resta agli italiani se si subordinano i diritti alle contabilità di bilancio. I diritti sociali devono essere sempre garantiti e non degradati a meri limiti. Siamo consapevoli che occorrono severi controlli e che una spesa sbagliata deruba il cittadino. Ma attraverso una trappola mortalmente rigorista si può anche commettere lo stesso ignobile furto, impedendo la spesa pubblica solidale. La dimensione dei diritti è fondativa e fragilissima. È una dimensione che ha sempre bisogno di venir argomentata e difesa, tanto più in un periodo di grave crisi economica e politica come quello che stiamo vivendo. Noi del Movimento ricordiamo costantemente che i diritti potrebbero rappresentare una straordinaria opportunità di rilancio per la politica; un'occasione per riacquistare legittimità e incisività, tornando a occuparsi delle vite delle persone, dei loro corpi, delle loro esigenze e aspirazioni quotidiane; opportunità che finora, però, la vostra politica non ha colto. infine ricordare quell'accorato appello dei premi Nobel dell'economia contro il pareggio di bilancio in Costituzione, il quale recitava con forza che nessun Paese importante ostacola la propria economia con il vincolo del pareggio di bilancio. Per questo motivo non c'era e non c'è ancora oggi alcuna necessità di far indossare al nostro Paese una camicia di forza economica come quella che è stata voluta da Monti, e non solo da Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, quello al nostro esame è un disegno di legge che riguarda la contabilizzazione delle poste di bilancio delle Regioni e degli enti territoriali; prevede la correzione della legge rinforzata di attuazione della norma costituzionale sull'equilibrio di bilancio, adottata dopo la modifica - avvenuta nel 2012 - dell'articolo 81 della Carta fondamentale e si pone come obiettivo primario utilizzare in modo più appropriato le risorse di cui dispone ogni singolo ente preposto al governo del territorio. La legge rinforzata viene sottoposta, per così dire, a un "tagliando". Infatti, questa revisione ci vedrà impegnati sia su questo provvedimento, che riguarda gli enti territoriali, che sul disegno di legge approvato dalla Camera e ora all'esame della

Gli obblighi europei, la legge costituzionale e poi la legge rinforzata, che - lo hanno già ricordato i colleghi - è una legge ordinaria molto particolare, in virtù della maggioranza assoluta necessaria per la sua approvazione, hanno posto precisi vincoli agli equilibri di bilancio. Ora si prevede che i bilanci degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, Province, Città metropolitane e Comuni) siano da considerare in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che in quella di rendiconto. Si riducono, quindi, i vincoli sui bilanci, ma rimane, comunque, un controllo preventivo e consuntivo sul saldo finale di competenza. Viene previsto che il fondo pluriennale vincolato, destinato alle spese in conto capitale, possa facilitare la programmazione delle spese sul territorio, favorendone un'integrazione, che porti a un livello maggiore di investimenti. Per gli enti del territorio si manifesta la possibilità di riclassificare l'eventuale indebitamento in quote costanti, divise in tre anni. Va registrato anche il tentativo di un cambio di mentalità, in questo disegno di legge, nel modo di affrontare i problemi dei livelli di governo del territorio, perché, finalmente, nei confronti degli enti del territorio vengono introdotti anche dei premi e non solamente delle sanzioni, come è stato finora, tra l'altro con un meccanismo apprezzabile come quello inserito durante i lavori della Commissione bilancio. Probabilmente si è preso atto che i livelli di governo più vicini alla gente hanno subito troppe penalizzazioni e sono quelli che negli ultimi anni hanno pagato il prezzo più alto all'equilibrio dei conti pubblici. Troppi sono stati i sacrifici immolati in nome dei saldi di bilancio e troppe le coperture finanziarie ricavate attraverso tagli ai trasferimenti a Comuni, Province e Regioni, utilizzate in sede di leggi di spesa, fossero esse leggi finanziarie o uno dei tanti decreti legge nati con l'intento di "salvare" l'Italia. Sbagliata si è rivelata anche l'idea di utilizzare lo strumento dell'imposizione fiscale comunale per destinarla - per oltre il 40 per cento delle risorse complessive - alla perequazione orizzontale nei confronti degli altri enti locali. Va sottolineato, inoltre, che le sole regole relative al Patto di stabilità interno e alla nuova contabilità hanno prodotto tagli sui bilanci comunali per oltre 3 miliardi di euro nell'ultimo quinquennio. La realtà è che i cittadini non possono davvero fare a meno dei servizi resi sul territorio alla collettività, perché sono quelli materialmente più vicini ai loro bisogni. Il sacrificio - voglio ricordarlo - è stato pesante, riuscendo a ridurre le risorse totali a disposizione dei Comuni (scese negli ultimi cinque negli 8.000 Comuni) e ad abbattere il volume degli investimenti sui loro territori (calati del 25 per cento nello stesso periodo). Le Province, con le poche risorse rimaste, non riescono nemmeno a far fronte alle funzioni essenziali individuate dalla legge Delrio, che, sostanzialmente, le ha svuotate di competenze. Ma, tra queste competenze ce ne sono - ad esempio - due sulle quali il taglio ha un impatto importante. Il primo esempio che vorrei fare è la manutenzione delle strade: vediamo ogni giorno, nelle nostre come è ridotto il manto delle strade controllate (130.000 chilometri di competenza). Il secondo esempio riguarda le scuole superiori: 5.000 in tutta Italia, sempre più fatiscenti, dove l'allarme per i crolli di intonaci o controsoffitti è ricorrente. Ed è veramente triste pensare che anche la solidità di un edificio scolastico è diventata uno dei parametri da considerare per la scelta della scuola da fare frequentare ai nostri figli. Come è altrettanto triste pensare che i genitori debbano provvedere ad autotassarsi per comprare beni di primaria utilità. Ebbene, a causa dei tagli, quest'anno le Province registreranno un disavanzo strutturale di oltre un miliardo di euro. Persino le Regioni, la cui funzione fondamentale dovrebbe essere quella di garantire *standard* di servizi qualitativamente omogenei, come - ad esempio - nel primario settore della sanità, continuano ad avere dei bilanci in sofferenza. Sappiamo tutti che, purtroppo, anche loro hanno pagato un prezzo importante in nome delle manovre di finanza pubblica. Le stesse Regioni ora vivono in un limbo sino alla celebrazione del *referendum* costituzionale che, qualora venisse approvato, le relegherebbe a competenze marginali, essendo stata ridotta - come sappiamo - la loro potestà in conseguenza della riscrittura del Titolo V della Costituzione. Al contrario, servono risorse economiche e, sopratutto, è necessaria una programmazione pluriennale della spesa che faccia ripartire gli investimenti. È ormai fondamentale la creazione di un nuovo quadro di finanza pubblica locale che coinvolga e responsabilizzi pienamente tutti i livelli di governo del territorio. tornare a un quadro di risorse proprie che possa garantire un livello di entrate tale da assicurare i livelli essenziali dei servizi e delle prestazioni resi su ciascun territorio. In cambio, lo Stato deve però ridurre il peso del prelievo fiscale centrale. Al contrario, leggiamo che gli unici dati certamente positivi che arrivano sull'operato di questo Governo sono quelli relativi all'andamento delle entrate, che registrano le tasse a carico degli italiani in continuo aumento, nonostante il sostanziale stallo del PIL. Purtroppo, anche la nuova articolazione delle leggi di contabilità che riguardano gli enti territoriali fa permanere quella incertezza dovuta a un quadro di programmazione annuale (quindi basato su un periodo troppo breve), che dipende dalle leggi annuali di bilancio e dalle conseguenti scelte di finanza derivata. in questo momento, essa risente anche degli errori nelle scelte di politica economica commessi negli ultimi anni e delle troppe cambiali. Mi riferisco alle clausole di salvaguardia su IVA e accise, che il Governo ha deciso di far gravare sui conti pubblici per i prossimi anni.

2012, n. 243, intende conseguire una pluralità di finalità. In primo luogo, esso cerca di operare un importante intervento di cui hanno molto hanno molto bisogno gli enti locali e le Regioni. Mi riferisco alla semplificazione del quadro normativo relativo al tema dell'equilibrio di bilancio. Con riferimento agli ambiti che riguardano gli enti decentrati come Regioni ed enti locali, invece, il provvedimento intende garantire e semplificare la possibilità per gli stessi enti di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali favorendo in tal modo una politica espansiva. Sappiamo tutti che di questo noi abbiamo molto bisogno e che, per sostenere la ripresa, sono necessari investimenti

di tetti alle spese che ha spesso impedito che gli investimenti si facessero anche laddove c'erano le risorse necessarie. Per troppi anni abbiamo avuto un sistema che ha

corroborata, la necessità di un rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture sia immateriali che materiali. Il disegno di legge che siamo chiamati a esaminare è finalizzato all'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, rafforzando il ruolo delle Regioni quali cabine

non toccando le disposizioni che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla Le modifiche si appuntano su tre specifici aspetti e intervengono sui commi 3, 4 e 5 e dell'articolo 10 della suddetta legge n. In particolare, la prima modifica stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima amministrazione regionale. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale. Con la seconda modifica si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243, con il quale si prevede in sede di rendiconto, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo nel complesso degli enti della Regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dalle modifiche introdotte che non prevedono più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. Infine, la modifica al comma 5 dell'articolo 10 ridefinisce, precisandola, la disciplina relativa ai criteri e alle modalità di attuazione del summenzionato articolo. del Consiglio dei ministri e prevede che siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e Province autonome. Dunque, nel complesso, si tratta di un provvedimento che intende, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio, favorire la capacità di investimenti sul territorio attraverso sia il ricorso al debito che l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle Regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento di ogni singola Regione. un provvedimento importante, che semplifica e agevola il lavoro fondamentale del sistema degli enti locali e delle migliaia di sindaci e centinaia di consiglieri e amministratori regionali che spesso sono troppo vincolati nel loro lavoro. Esso determina le condizioni per un intervento più sostenuto sul fronte degli investimenti per sostenere una ripresa che i provvedimenti del Governo nel nostro Paese e il rapporto che ormai abbiamo stabilito in Europa con la flessibilità che siamo riusciti

prodotto alcune sollecitazioni cui provo a rispondere in modo sintetico, anche perché molti interventi hanno ripercorso un po' la storia del contenuto del documento e, soprattutto, la storia degli enti locali dal 2010-

dal 2014, ma in particolare nel 2015, molte cose sono cambiate per gli enti locali. È chiaro che ancora tanta strada è da fare, ma molto molto è cambiato. C'è stata sicuramente un'inversione di tendenza, sia nel decreto-legge n. 78 del 2015, sia nella legge di stabilità 2016 che, per la prima volta, anziché

Alcune osservazioni della Corte dei conti sono addirittura di maggior attenzione: se volessimo davvero guardare al documento prodotto nel corso delle audizioni,

terrà conto delle nuove normative sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e sarà quella la prima sede in cui si comincerà a parlare nuovamente di finanziamenti. Infatti, torno a ripetere,

e un processo di ricollocazione del personale che è stato sicuramente il più grande dal dopoguerra ad oggi, perché il numero delle persone da ricollocare era davvero elevato.

non si lamentavano affatto, perché dal fondo di solidarietà comunale avevano avuto una grossa entrata. Quindi quelli che si vedevano ridotta l'entrata strillavano molto, ma gli altri stavano in silenzio, belli coperti, per non entrare troppo in discussione.

e comunque il processo che è stato attivato è sicuramente un processo virtuoso, che aiuterà a cominciare a scrivere i bilanci per il 2017 in tempi utili. Il pezzetto che facciamo oggi è sicuramente un tassello di questo*puzzle* ed è un tassello molto importante.

il confronto in Commissione bilancio sulla riforma della legge n. 243 del 2012 si è svolto in un clima di autentica collaborazione tra i Gruppi.

così come definito dalla legge n. 243) sono stati presentati gli stessi emendamenti con le firme dei senatori di maggioranza e dei senatori di opposizione, a dimostrazione, al di là del disegno di legge del Governo, di un comune sentire che c'è tra le forze politiche sulla questione della decisione di bilancio e della tenuta del bilancio degli enti locali e delle Regioni.

la realtà si incaricherà di dimostrarlo - con il fatto che ormai tutte le principali forze politiche del Paese, in questo piuttosto che in quell'altro Comune, sono chiamate a svolgere funzioni di Governo e quindi si pongono il problema della decisione di bilancio e della corretta gestione del bilancio degli enti locali come un problema di tipo trasversale alle forze politiche. Ora, è bene che sia così perché queste due norme, quella contenuta nella legge di contabilità, giunta al Senato dalla Camera, e quella che ora ci apprestiamo ad esaminare in Aula qui al Senato, relativa alla legge n. come si dice in gergo, norme di sistema, cioè norme che hanno rilievo costituzionale (anche se non sono legge costituzionale), perché la legge di contabilità e la legge cosiddetta rafforzata n. 243 sono entrambe essenziali per rendere possibile l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e, finché è in vigore, la Costituzione non è del Governo e delle maggioranze *pro tempore*: la Costituzione è la Costituzione. D'altra parte - ce lo ha insegnato la storia - i Parlamenti, come noi oggi li conosciamo, nascono sulla decisione di bilancio; nascono quando Giovanni Senzaterra, all'inizio del 1200, è costretto a concedere ai baroni inglesi, che stavano marciando su Londra perché si erano stufati di pagare guerre che non avevano contribuito a decidere, la Magna Charta Libertatum, in cui sostanzialmente il sovrano è costretto ad attribuire una forma di codecisione sul bilancio e sulla scelta di fare guerra, cioè sulla guerra e sul modo di finanziarla, da condividere con un'assemblea di rappresentanti. Non dico che quello fosse un Parlamento come oggi lo conosciamo, ma è significativo che il principio fondamentale, e cioè nessuna tassazione senza rappresentanza e nessuna rappresentanza senza una qualche forma di partecipazione a contribuire alle spese dello Stato attraverso la tassazione, abbia secoli di storia dietro di sé. Quindi quella di bilancio è una decisione costituente per i Parlamenti,

c'è, al di là del fatto che adesso in Aula si ricorra sempre a qualche elemento polemico, che è pienamente giustificato dal fatto che ci si rivolge da questi banchi anche direttamente al Paese. Vi garantisco che in Commissione niente di tutto ciò è accaduto e c'è stata una discussione sul merito. Venendo al merito, perché è necessaria la riforma della legge n. per la parte di quella legge che riguarda il bilancio delle Regioni e delle autonomie locali? Per rispondere correttamente, bisogna tornare all'articolo 81 della Costituzione,

se faccio il pareggio sia in condizioni di crescita particolarmente intensa sia in condizioni di recessione, sto negando alla politica fiscale di bilancio la possibilità di intervenire, quando c'è crescita particolarmente intensa, attraverso l'avanzo per "mettere in cascina" le risorse necessarie per intervenire quando la recessione suggerirà di attuare politiche in disavanzo. la questione è molto semplice: ma è fondato il giudizio che si dà sull'articolo 81 così come è scritto in Costituzione? È evidente che questo giudizio non è fondato, perché l'articolo 81 della Costituzione afferma il principio dell'equilibrio di bilancio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico».

del senatore Buccarella).* Mai in Costituzione si sarebbe potuto fare uso di una nozione tecnica come quella di pareggio strutturale, quindi il costituente ha scritto l'equilibrio di bilancio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Questo cosa vuol dire? Che il vincolo non è costituito dal pareggio nominale di bilancio. Il pareggio nominale di bilancio è:

del saldo di bilancio. Quando il Paese è in recessione si tratterà di una oscillazione verso il basso, cioè verso l'indebitamento, per consentire politiche fiscali anticicliche, è questa la novità - che quando non c'è recessione, anzi quando c'è crescita appena significativa, naturalmente il bilancio vada in avanzo, al fine di oscillare attorno allo zero finanziando le fasi nelle quali, invece, bisogna fare disavanzo. Questo è il principio fissato in Costituzione. Uno può essere favorevole a questo, oppure contrario, può proporsi, programmaticamente, di modificare

il vincolo del pareggio di bilancio nominale, cosa palesemente non vera. Tant'è, l'articolo 81 della Costituzione dice che «Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo Perché mai si sarebbe scritto in Costituzione che il ricorso all'indebitamento è consentito quando il ciclo economico imponga di considerare il suo carattere negativo, se l'obiettivo fosse il pareggio nominale? Non avrebbe senso questa norma in Costituzione, se le cose non stessero esattamente come ho cercato

laddove naturalmente esso è fissato, oggi, dalla legge n. 243 (esattamente la legge di cui stiamo discutendo, esattamente nella parte di cui ci stiamo occupando con una proposta di modifica), con la previsione dei famosi quattro saldi: bilancio di previsione, bilancio di rendiconto, pareggio di bilancio pareggio di bilancio sul versante della competenza e della cassa, sul versante delle entrate e delle spese correnti. Un obiettivo fissato in termini talmente rigidi da rendere, a mio avviso, necessario un intervento correttivo. La ragione per cui siamo qui è questa: introdurre un correttivo nella tenuta dei bilanci degli enti, delle Regioni e dei Comuni, in modo tale da superare l'eccesso di rigidità

competenza tra entrate finali e spese finali deve essere in pareggio. Naturalmente, interveniamo di conseguenza su quella parte della

di introdurre il principio della politica fiscale anticiclica anche per quanto riguarda gli enti locali, con ciò naturalmente determinando un complesso di norme che, incrociandosi tra di loro, apparivano eccessivamente rigide. eccessivamente rigide. Nella Commissione bilancio abbiamo ulteriormente sviluppato la modifica già proposta dal Governo su questa parte per introdurre, attorno al fondo di solidarietà, il principio secondo il quale, attraverso politiche fiscali decise nazionalmente, lo Stato può consentire al sistema delle autonomie locali, con maggiore facilità e sulla base del principio della corresponsabilità degli enti locali di ciascuna Regione (compresa la Regione), lo sviluppo di politiche anticicliche quando il ciclo sia negativo.

a proposito della decisione di bilancio e delle caratteristiche della politica di bilancio degli enti locali, che rispondesse all'esigenza di maggiore flessibilità in in un contesto nel quale era fissato e veniva ribadito il principio del pareggio di bilancio, nel caso nel caso degli enti locali, di tipo nominale e non strutturale, ricorrendo, per la caratterizzazione del pareggio strutturale del bilancio degli enti locali, al meccanismo del concorso dello Stato centrale. Questo contesto è largamente condiviso

le soluzioni, almeno in parte, divergevano: un problema molto importante. Voi sapete che, per quello che riguarda la tenuta dei bilanci del 2016, con legge di stabilità il Governo ha proposto - e il Parlamento ha ulteriormente allargato allargato - gli spazi per la finanza degli enti locali, in particolare sul versante dell'utilizzo, attraverso la creazione del fondo pluriennale vincolato, di quote di avanzo di amministrazione che il carattere - questo, sì, stupido - del Patto di stabilità interno, degli ultimi quasi vent'anni, aveva finito per gonfiare. È ovvio, infatti, che se si stabilisce un Patto di stabilità interno che impone l'avanzo che impone l'avanzo ai bilanci degli enti locali, nel tempo, di avanzo in avanzo, si costruirà un gigantesco avanzo degli enti locali.

ha ragione, tant'è vero che su questo c'è la svolta 2016: almeno in parte, con il fondo pluriennale vincolato, quote dell'avanzo entrano nella possibilità di essere utilizzate, in particolare per la spesa in conto capitale.

si decide quanto e come del fondo pluriennale vincolato entra nel saldo. La soluzione proposta dalla relatrice e poi approvata dalla Commissione rovescia questo principio e dice esattamente il contrario, venendo così incontro a una sollecitazione che viene dal sistema delle autonomie, governato da chiunque sia, da tutti: dice che il fondo pluriennale vincolato è componente del saldo. A regime è così, punto a capo. Ciò accade dal 2020 e attenzione a pensare che su argomenti di questo tipo il 2020 sia particolarmente lontano. affermando che tra il 2017 e il 2019, non la legge annuale - come diceva originariamente il Governo - ma la legge triennale di bilancio stabilisce le regole attraverso le quasi il fondo pluriennale vincolato entra nel saldo.

mese, ma in una norma di sistema l'essenziale è avere stabilito che il fondo pluriennale vincolato è dentro il saldo e lo è dal 2020. Questo è un vero salto di qualità ed emendamenti per ottenere tale risultato erano stati presentati da tutti. Visto che lo avete ottenuto, tenderei a sottolineare il fatto positivo piuttosto che la differenza sulla soluzione nella transizione tra il 2017 e il 2019.

salvo vedere come regolare la fase di transizione verso il conseguimento di quella soluzione a regime. Ho concluso il mio intervento; ringrazio la relatrice e tutti non c'è dubbio che il provvedimento che viene portato in Aula per l'approvazione è decisamente diverso, su un punto fondamentale, da quello proposto originariamente dal Governo e secondo me è una diversità lo dice il Governo così credo lo possano condividere tutti - positiva e non negativa.

dell'istituto penitenziario di Monza. Avevo presentato tale interrogazione dopo una serie di eventi che avevano coinvolto il personale in qualche episodio assolutamente spiacevole e pericoloso, sia per i detenuti che per le guardie di Polizia penitenziaria. A seguito della mia interrogazione sono andato a sincerarmi personalmente della situazione in cui versa il carcere di Monza e ne ho tratto alcune considerazioni

la necessità di dotare queste carceri, in particolare quello di Monza, della possibilità di coinvolgere davvero i detenuti in un processo di riabilitazione che li veda protagonisti anche di qualche attività sportiva. In questo senso, mi è stata segnalata una grande

Signora Presidente, purtroppo un ennesimo omicidio si è consumato tra le mura domestiche. Questa volta è successo in un appartamento alla periferia di Torino, dove una donna è stata trovata in casa senza vita. La donna, Diana Gogoroia, moldava di trentasei anni, da tempo residente in Italia, è stata trovata nel letto con la gola tagliata, mentre il suo convivente Antonio Missud, un italiano cinquantunenne con precedenti per minaccia e violenza alle persone, è stato trovato in una stanza vicina, impiccato. Gli inquirenti ritengono che si possa trattare di un omicidio-suicidio con al centro il fattore gelosia. La donna era appena rientrata da un viaggio che aveva effettuato da sola per qualche settimana. Da quando è iniziata la staffetta che abbiamo deciso di effettuare qui in Senato, giorni fa, sono già quattro le donne uccise per mano di un uomo cui erano legate da relazione sentimentale. Con questo intervento continua oggi la staffetta con cui, assieme ad altre senatrici, ricorderemo ogni donna che verrà uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna, e il 46 per cento di queste donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata e sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Sui *media* la violenza sulle donne è quasi sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'onore tradito, che giustificava il delitto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare: il suo è stato un gesto estremo. Una spiegazione, insomma, che, dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità, in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano, per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Sul caso di Diana Gogoroia, che cosa non ha funzionato? Il suo convivente aveva precedenti per minacce e violenza alle persone. Ci domandiamo, allora ripetere tre appelli. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto, affinché si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al Piano d'azione Un appello ai *media*, affinché si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne e si contribuisca alla crescita della cultura del rispetto di tutte le donne e di tutte le persone. Infine, un appello al Paese, agli uomini e alle donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, forse non avete avuto modo di conoscere la notizia attraverso gli organi di stampa nazionali, perché non fa molto clamore, ma colgo l'occasione per aggiornarvi sul fatto che nella città di Ventimiglia la pressione del flusso migratorio di persone provenienti dall'Africa subsahariana, in particolare dalla Nigeria, dall'Eritrea e dal Sudan, sta mettendo seriamente in crisi le scarse disponibilità di risorse delle associazioni caritatevoli, in particolare la Caritas, che in questo momento stanno supplendo all'intervento all'intervento dello Stato, in attesa dell'apertura di un campo per l'accoglienza - per fornire informazioni sulla possibilità di richiesta di asilo o di protezione internazionale e il primo soccorso - che avverrà nei prossimi giorni presso l'area del Parco Roja. Le presenze odierne sono state quantificate in circa 1.200 persone, molte delle quali sono arrivate nel nostro Paese attraverso i famigerati viaggi della morte sui barconi, spesso tramite la rotta egiziana. Molte di loro probabilmente sono già state identificate presso le diverse strutture nel Sud Italia e non è la prima volta che tentano di valicare i nostri confini nazionali, al fine di raggiungere altri Paesi europei. L'estate scorsa, con l'intensificarsi dei controlli al confine francese, si arrivò a un picco di 800 persone ferme sul territorio ventimigliese, circa un centinaio nelle immediate vicinanze del confine di

grandissima solidarietà dimostrata dai cittadini ventimigliesi, che immediatamente accorsero in aiuto, portando indumenti, coperte e generi di prima necessità. Quest'anno, con l'avvicinarsi dell'estate, il flusso migratorio è ripreso e, nel mese di maggio, circa duecento migranti si accamparono alla foce del fiume Roja, successivamente ricevettero ospitalità nelle chiese della diocesi di Ventimiglia, ma a giugno, tra le riammissioni sul suolo italiano da parte delle autorità francesi, che hanno proceduto a un ritmo di circa 50 persone al giorno in media, e gli arrivi dal Sud Italia, il numero delle persone ospitate nella chiesa di sant'Antonio, nel quartiere delle Gianchette, ha continuato a crescere, nonostante la forte mobilità dei migranti stessi, fino a raggiungere l'attuale numero di 1.200 persone. Il Ministero dell'interno ha provveduto con controlli nelle stazioni di Genova e Savona a costituire dei "filtri" che impedissero l'arrivo dei migranti nella città di confine e, tramite la Prefettura, in concerto con l'amministrazione comunale ventimigliese, sta procedendo all'allestimento

fortuna nell'antistante posteggio e nuovamente sulle rive del fiume Roja, con a disposizione solo due servizi igienici. Capite che il sistema idrico e fognario rischia il collasso, con conseguenze gravi sul piano sanitario. Un'altra questione che merita attenzione è la crescente tensione sociale. La città di Ventimiglia e le associazioni di volontariato stanno facendo il possibile, ma da soli non possono dare risposte efficaci ai migranti e agli abitanti del quartiere. Vorrei sottolineare anche gli episodi di strumentalizzazione politica xenofoba, che tendono a fomentare tali tensioni, in particolare della Lega Nord, anche se diverse organizzazioni della destra extraparlamentare non sono da meno. La situazione ventimigliese merita attenzione, a tutela dei cittadini e dei migranti. Sarete anche a conoscenza del triste fenomeno dei *passeur*, sciacalli che, dietro pagamento, promettono il valico del confine ai migranti tramite sentieri o tramite il loro trasporto su mezzi come furgoni o camion. Fortunatamente non si sono verificate tragedie come quella austriaca dell'estate scorsa, quando 71 migranti furono trovati morti asfissiati dentro un camion abbandonato, ma il rischio è quello. Senza contare che la criminalità organizzata potrebbe trovare terreno fertile anche nella tratta - perché di questo stiamo parlando - dei migranti, dal momento che la presenza della 'ndrangheta nel Ponente ligure è ribadita dalle sentenze del processo La Svolta. Gentili colleghi, vi chiedo di sostenere presso le sedi istituzionali ogni possibile aiuto che possa allentare tale tensione sulla città di Ventimiglia e chiedo al Governo di concordare con l'amministrazione comunale, la questura locale e le organizzazioni umanitarie maggiori risorse e maggiori spazi per l'accoglienza dei migranti, nonché maggiori strumenti informativi presso gli stessi. Concludo infine con un auspicio a riguardo della protezione dei minori non accompagnati. È notizia recente la volontà del Governo di raddoppiare il fondo dedicato e di aumentare gli sgravi a carico dei Comuni ospitanti i piccoli migranti. Vi prego: date nel più breve tempo possibile attuazione a tale volontà. Non è possibile che molti bambini cadano ancora nelle mani di chi intende sfruttarli e che di molti di loro se ne perdano le tracce. L'Italia è un Paese che accoglie, è un Paese che rispetta e attua la legislazione internazionale ed europea per quanto concerne il rispetto dei diritti umani. L'Italia non deve permettere che a Ventimiglia questo non possa avvenire.

Ben 21 milioni di italiani praticamente lo usano ogni giorno! Un servizio di rete sociale - così loro si definiscono - decide improvvisamente, in modo del tutto arbitrario, che un documentario di nazionalità italiana con normale visto di censura e divieto ai che ha rappresentato il nostro Paese in festival internazionali come i festival di Rotterdam, Buenos Aires, Varsavia, San Paolo, e Mosca, proiettato un paio di settimane fa in uno dei luoghi simboli del cinema francese a Parigi, al Forum des images a Les Halles - debba essere oscurato, censurato e tolto dalla circolazione. Perché, chiederete? Perché il manifesto di questo documentario, caricato sulla pagina ufficiale di Facebook, mostra un capezzolo (che peraltro compare in una scena tratta da un film del 1970 usata come locandina). Il capezzolo di una donna secondo gli *standard* di Facebook è poco "rispettabile". Ma la cosa ancora più grave è che Facebook questa volta non si è limitato soltanto a censurare un'immagine, così come aveva già fatto per il famoso dipinto di Courbet, «L'origine du monde». In questo caso, infatti, il *social network*, senza nessuna spiegazione ufficiale, senza un preavviso e senza aver mai risposto alle richieste di spiegazioni da parte degli autori del documentario, oscura e fa sparire la stessa pagina che promuoveva il film, frutto di un lavoro costruito in un anno e mezzo con migliaia di utenti.

Facebook non solo si fa censore, ma infligge anche sanzioni senza possibilità di replica, come in un processo sommario dove manca la possibilità di difendersi. Si tratta di una vera e propria violazione della libertà di espressione, di una grave ingiustizia per un film indipendente nato anche grazie al sostegno della rete. Giova, inoltre, sottolineare come l'elemento il documentario in questione racconti la storia di un gruppo di persone che cinquant'anni fa, in un'Italia iper-religiosa, democristiana e bigotta e con un Partito Comunista ancora più moralista, con grande coraggio e ostinazione, subendo ogni sorta di linciaggio, hanno lottato proprio contro la censura, per i diritti civili e la libertà sessuale. Sono persone che hanno subito condanne e che sono state arrestate anche affinché il seno di una donna potesse essere visto alla luce del sole e fotografato senza essere censurato. Ahimè, un film contro la censura viene censurato. si lasci infine lamentare a gran voce il silenzio istituzionale assoluto in merito (oggi mi informo). Per quanto attiene ad opere intellettuali interamente concepite in Italia non sembra giusto che l'autorità censoria sia interamente di competenza di soggetti stranieri. Non è accettabile che alcuna voce in merito si levi dai Governi statali interessati, Governi di Paesi che - lo si diceva - hanno superato con dure lotte le strette strette maglie della censura e che dovrebbero essere in prima linea a difendere quei diritti civili così duramente conquistati anche contro imprenditori stranieri che paiono essere storicamente molto indietro su questi temi.

Presidente, 40 lavoratori del cantiere NCA di Marina di Carrara lanciano in questi giorni un appello e chiedono aiuto ai politici onesti e ai cittadini, aggiungendo aggiungendo che se l'azienda crede che il denaro sia la medicina per tutto loro rispondono che il lavoro non si compra e non si vende. Presidente, sposo appieno il loro appello e non solo: aggiungo se ancora siamo in uno Stato di diritto e non in uno Stato di regime, ho il diritto ad avere risposte alle mie numerose interrogazioni presentate riguardo - mi si lasci passare il termine - le schifezze che si stanno facendo sulla pelle dei lavoratori del cantiere NCA di Marina ora di smettere di fare orecchie da mercante. Presidente, il primo atto l'ho depositato all'attenzione del ministro Poletti il 17 febbraio 2015, il secondo l'avevo rivolto all'ex ministro Guidi il 22 aprile 2015, gli interventi in Aula sul tema NCA ormai non li conto più. Un'altra interpellanza la depositai il 30 novembre 2015, con procedura abbreviata nella speranza di avere risposta: tutto inutile. Adesso sul caso NCA e del Porto di Carrara sta anche indagando la procura, sul caso del reinserimento lavorativo di operai e impiegati in cambio di molte concessioni, tra cui quella demaniale per trent'anni con scadenza il 31 dicembre 2042. La procura, come sempre, arriva prima dei politici e prima del Governo? del Governo? In questa faccenda sono coinvolti molti protagonisti. Non vorrei dover pensare che qualcuno sia considerato, in questo vergognoso caso, un intoccabile. Presidente, la rabbia dei lavoratori che stanno rischiando il licenziamento è la mia stessa rabbia. L'indignazione per l'abbandono totale delle parti, come detto da loro, istituzionali, sindacali e territoriali è la mia stessa indignazione. Oggi ho pronta una quarta interrogazione che arriverà nuovamente nei cassetti di vari Ministri. Cosa devo fare, come parlamentare e rappresentante del popolo per farmi considerare, Presidente, mi devo dare fuoco? Quello che sta avvenendo a Marina di Carrara è gravissimo e poteva essere evitato. Sono più di due anni che il Movimento 5 Stelle si sta battendo affinché venga fatta chiarezza sul caso NCA. Nelle mie interrogazioni chiedo anche accesso a dati e documenti che costituiscono parte integrante dell'accordo che ha permesso la cessione della società controllata da Invitalia ad un privato, l'imprenditore Giovanni Costantino, con patto di reinserimento dei lavoratori. Quindi, come dicevo, aspettiamo ancora i comodi dei vari Ministeri o cominciamo cominciamo a pensare che la procura ci debba fornire i dati di cui abbiamo bisogno? Presidente, pochi giorni fa ho incontrato nuovamente i lavoratori della società NCA e tendo a ribadire il concetto che la dignità non ha prezzo prezzo e che non tutti sono ancora in vendita. Fintanto che il lavoro sarà un nostro diritto, sancito dalla Costituzione e inserito addirittura nel suo primo articolo, noi del Movimento 5 Stelle saremo al loro fianco e lotteremo con loro per ottenere risposte e giustizia.